finestra") ***Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti***

il decreto n. 61 che ci accingiamo a convertire in legge, recante interventi straordinari per superare l'emergenza rifiuti in Campania, riconferma lo sforzo che il Governo sta compiendo, attraverso il commissario delegato, per porre fine a un'intollerabile situazione di degrado ambientale e sociale che impropriamente va sotto il nome di emergenza rifiuti e che da troppo tempo si protrae, con pesanti ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini della Regione. Sulla conversione in legge del decreto n. 61 si è svolto in Commissione un approfondito dibattito, al quale hanno dato il loro importante contributo tutti i commissari di maggioranza e di opposizione, e di ciò voglio qui ringraziarli in maniera assolutamente non rituale. La Commissione ha anche avuto modo di svolgere una serie di audizioni (in particolare di rappresentanti della struttura commissariale, dei presidenti delle Province campane, dei sindaci dei Comuni individuati all'articolo 1 del decreto, del presidente della Federparchi, del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente), che hanno ad essa consentito sia di mettere a fuoco alcuni specifici aspetti della realtà effettuale e istituzionale, sulla quale la normativa del decreto va ad incidere, sia di disporre di una visione di insieme dell'attuale situazione emergenziale, nonché delle sue prospettive di evoluzione, con particolare riferimento al percorso che dovrà da qui alla fine dell'anno portare al passaggio all'ordinarietà nella gestione del ciclo dei rifiuti. In effetti*,* quello che il Presidente della Repubblica ha definito il penoso protrarsi dell'emergenza rifiuti in Campania ha ormai, a distanza di 14 anni dalla nomina del primo dei sei commissari straordinari, tutte le caratteristiche di una condizione cronica inaccettabile, priva di qualsiasi giustificazione e segnata in più punti da responsabilità specifiche e diffuse, da responsabilità locali e da sottovalutazioni istituzionali anche nazionali. Errori strategici e gravi inadempienze hanno condizionato le scelte di questi 14 anni, con il risultato che sovente il ricorso a interventi per l'emergenza ha prodotto nuova emergenza. A tutt'oggi, si deve ancora chiudere il ciclo dei rifiuti, non solo nel senso di superare definitivamente l'emergenza ma soprattutto nel pervenire alla realizzazione di un ciclo integrato nel quale ogni componente faccia la sua parte. A tutt'oggi è forte la consapevolezza che il successo di questa intrapresa è anche legato alla capacità di resistere a quelle penetrazioni e a quei condizionamenti della criminalità organizzata che purtroppo in tutti questi anni hanno segnato e influenzato l'emergenza rifiuti in Campania. Dunque, la gravità della situazione esige ancora oggi interventi di tipo straordinario, anche per rimuovere con assoluta celerità condizioni ambientali suscettibili di produrre nuovi effetti negativi sulla salute delle persone, ma esige altresì che la condizione di un piano di gestione integrata del ciclo dei rifiuti si ponga come condizione necessaria per chiudere l'emergenza e per superare in modo realmente definitivo l'attuale situazione di degrado. Giustamente, pertanto, il decreto-legge in conversione salda il riconoscimento di ampi poteri al commissario delegato - nella linea già tracciata dal decreto n. 263 del 2006 - con la previsione, all'articolo 9, di un piano per il ritorno all'ordinarietà e con la nomina, all'articolo 6, dei Presidenti delle Province a subcommissari al fine di accelerare la restituzione dei poteri agli enti competenti. Quest'ultima previsione va collegata a quella, sempre all'articolo 6, secondo la quale il Presidente del Consiglio, su proposta del commissario, revoca lo stato di emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali in possesso di sufficiente dotazione impiantistica. Siamo qui di fronte a uno dei profili cruciali del decreto: l'urgenza di taluni straordinari interventi e il relativo accentramento di competenze sono correlati e preordinati all'instaurazione dell'ordinarietà. Peraltro, sull'ordinarietà non vi è nulla da inventare in Campania; esiste un quadro legislativo sia nel nostro Paese che a livello europeo, che, laddove è stato attuato, ha prodotto - e questo vale anche per buona parte delle Regioni italiane risultati importanti in termini di condivisione e di efficienza del ciclo integrato dei rifiuti, capace non solo di allontanare l'emergenza, ma di rendere possibili, oggi, frontiere ancora più impegnative sul terreno della riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata e del riuso del materiale riciclato. Il dibattito svoltosi in Commissione ha evidenziato queste tematiche e soprattutto è valso a mettere in rilievo come questo piano, se vuole davvero segnare la chiusura dell'epoca non gloriosa dell'emergenza, deve essere un piano condiviso, un piano che nasca dalla comunicazione e dal dialogo responsabile con le istituzioni locali e con i cittadini, secondo quella logica di partecipazione e di informazione che ha caratterizzato che ha caratterizzato il decreto-legge n. 263 del 2006 e che mantiene tuttora piena validità, anzi, oggi è ancora più valida di ieri. Il combinato disposto, previsto da questo decreto, tra affidamenti impegnativi al commissario delegato per l'oggi e un piano chiaro, credibile, possibile da avviarsi contestualmente alla fine dello stato di emergenza, è anche l'unica possibilità per recuperare credibilità e fiducia tra le istituzioni, ma soprattutto tra la popolazione della Campania, in particolare tra i cittadini di quelle località dove sono previste le realizzazioni indicate in questo decreto. decreto consta di 10 articoli. L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che entro il termine dello stato di emergenza rifiuti - fissato al 31 dicembre 2007 - sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti Comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. Il comma 2 consente l'utilizzo del sito di Serre fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della Provincia di Salerno. Il comma 3 consente l'uso del sito di Terzigno fino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa in esercizio del termovalorizzatore di Acerra. Sempre ai sensi del comma 3, il commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato esistenti nel medesimo territorio. L'articolo 2 disciplina l'affidamento del servizio di smaltimento e prevede che il commissario delegato individui, anche con affidamenti diretti, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti. Prevede altresì che il commissario delegato possa utilizzare, previa requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. L'articolo 3 vieta la localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell'area «Flegrea». L'articolo 4, al comma 1, obbliga i Comuni della Regione Campania ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della Regione Campania n. 10 del 1993. sensi del successivo comma 3, il commissario delegato può disporre l'accorpamento, ovvero lo scioglimento, dei consorzi medesimi che non adottino le misure che saranno prescritte da una specifica ordinanza commissariale, per l'incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata. L'articolo 5 stabilisce che i prefetti della Regione Campania, per quanto di competenza, assumano ogni necessaria determinazione per assicurare la piena effettività agli interventi e alle iniziative poste in essere dal commissario delegato.

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del commissario delegato, si possa provvedere alla revoca delle dichiarazioni dello stato di emergenza, anche limitatamente ai singoli ambiti provinciali che presentino sufficiente dotazione impiantistica. L'articolo 7 prevede che i Comuni campani debbano assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani garantisca complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio. I Consigli comunali che non provvedono nei termini previsti possono essere sciolti per grave violazione di legge. L'articolo 8 dispone che dall'attuazione del decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'articolo 9 stabilisce che, in sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il commissario delegato, entro 90 giorni adotta, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania e il commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione del ciclo industriale integrato dei rifiuti. signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, nel chiedere all'Aula l'approvazione della conversione in legge del decreto-legge n. 61, segnalo che la 13a Commissione ha approvato nel suo lavoro istruttorio, tenendo conto anche dei pareri delle altre Commissioni, alcuni emendamenti al testo originario che, senza intaccare in nulla le finalità del decreto, ne rafforzano, questo è l'intendimento, la praticabilità e l'incisività.

provvedimento, anche se non formalmente, configura sostanzialmente una reitera, prassi costituzionale ormai assolutamente censurata nell'attività dei Governi e quindi anche nella recettività da parte del Parlamento e dello stesso Presidente della Repubblica. Anche se dal punto

ad esaminare un decreto sulla cosiddetta emergenza rifiuti in Campania. Ma vi è di più. In questo decreto vi sono contenuti che aggravano ulteriormente le caratteristiche di incostituzionalità dello stesso. Mi riferisco, innanzitutto, all'individuazione di specifici siti che deriva dall'incapacità degli organi locali a trovare un momento di sintesi e di condivisione tre le varie amministrazioni e i vari livelli di governo locale,

anche con riferimento a pressioni di carattere politico e locale; addirittura, si fa intervenire il Capo dello Stato nel corso di una visita in Campania

però, che il compito di illustrare una questione pregiudiziale su questo decreto oggi è assai facile: basta scorrere i pareri delle Commissioni che hanno fornito il loro supporto a quella di merito. La 1ª Commissione permanente - anche se

destinati all'accoglimento e allo smaltimento dei rifiuti in aree di particolare valore paesaggistico e ambientale e già specificatamente protette a tal fine: sicuro, quindi, un principio costituzionalmente riconosciuto, quale quello della tutela dell'ambiente. Inoltre, vi è la situazione dei siti assoggettati a provvedimenti della magistratura per indagini penali,

Il parere della Commissione, infatti, è condizionato al fatto che alla previsione del possibile utilizzo di siti già sottoposti a sequestro vi sia un preventivo nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Questo, naturalmente, finisce per rendere vana la norma, entrando in perfetta contraddizione con la volontà del Governo, ma riallineerebbe dal punto di vista costituzionale la previsione. Ribadisco, di una previsione che, tra l'altro, infrange il principio, costituzionalmente riconosciuto, dell'autonomia e della separatezza dei poteri, ma - guarda caso - in una localizzazione ben camuffata. È chiaro, infatti, che un provvedimento di questo tipo può essere assunto solamente con il retropensiero di dover interessare certamente un sito già individuato e sequestrato dalla magistratura.

in maniera molto forte il contenuto dell'articolo 4, che prevede l'intervento sui cosiddetti consorzi di bacino,

consorzi già esistenti. Ciò entra pesantemente nell'autonomia dell'ente locale, costituendo, quindi, una palese violazione costituzionale, ai sensi del Titolo V della Costituzione.

delle prerogative regionali, con la possibilità dello scioglimento e dell'accorpamento dei consorzi. Quindi, la 1ª Commissione riesce ad arrampicarsi sugli specchi e addirittura - per giustificare le forzature costituzionali di questo decreto riferirsi all'articolo 120 della Costituzione, sulla tutela della salute pubblica (riferimento che potrebbe essere applicabile a qualsiasi intervento stravolgente l'assetto costituzionale e l'ordinamento dei nostri enti locali

come il decreto sia palesemente incostituzionale. Ripeto, l'incostituzionalità ancora più evidente è proprio,

anche sulla responsabilità degli enti locali. Abbiamo più volte richiamato la responsabilità soprattutto della Regione Campania e degli enti locali campani di non aver saputo affrontare adeguatamente questa vicenda. Oggi ancor di più con questo decreto li esentiamo da responsabilità di condivisione di quella gestione e, anche se ci sono dei pallidi tentativi di associarli non alle decisioni ma alle attuazioni attuazioni delle future decisioni del commissario delegato, certamente questo continua a configurare una palese intromissione indebita e incostituzionale sugli assetti

degli enti locali nella gestione della tassa per lo smaltimento rifiuti e ne impone una evidentissima lievitazione, anche se la 5a Commissione

approccio nella copertura dei provvedimenti del Governo e del Parlamento, qui si ha una sorta di inversione dell'onere della prova, nel senso che

non ci dice quanto costano quegli interventi in modo da poterne ricavare l'eventuale regolarità della copertura finanziaria, ma cita solamente la disponibilità

dal Tesoro, perché evitino, approvando la questione pregiudiziale, che si perpetri una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Dico ulteriormente approfondire - lo faremo certamente nel corso del dibattito - la palese violazione in ordine all'autonomia tributaria degli enti locali, che è pure materia sulla quale la 5a Commissione dovrebbe intervenire e per la verità è intervenuta con una piccola osservazione che vanifica assolutamente la previsione delle norme compensative a favore dei Comuni interessati e previsti dal decreto come oggetto dell'attività a loro carico che interessa l'intero territorio regionale. Quando le compensazioni a favore dei Comuni, per intervento della 5a Commissione, devono essere ricavate dalla tassa di smaltimento dei rifiuti imposta a tutti i cittadini, è evidente che il Governo si è voluto assolutamente tirare fuori dall'obbligo di dover intervenire in questa situazione di emergenza anche dal punto di vista economico e ha assolutamente vanificato la sua stessa norma, rendendola irridente. Così come ho suggerito - ne parleremo in discussione di merito - sarebbe molto più onesto da parte del Parlamento cassare completamente quella previsione che è palesemente inattuabile.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione le osservazioni svolte dal collega D'Alì per giustificare la mancanza dei presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge. In proposito devo dire, avvantaggiato dall'aver partecipato alla discussione sulla questione in Commissione affari costituzionali, molti degli argomenti che il collega ha trattato sono stati oggetto di un approfondito esame nella Commissione competente, che ha consentito di fugare qualsiasi dubbio e riportare gli elementi che sono stati tradotti poi in osservazioni in quel parere di cui pure ha dato alcun riferimento. Deve rassicurare il collega D'Alì e l'Assemblea che quel parere assolutamente positivo non è stato espresso soltanto per un dovere politico, né per una solidarietà

da ogni dubbio: la questione che ha posto in prima battuta il collega D'Alì, che è stata oggetto di una sentenza della Corte costituzionale del 1996 a proposito della non reiterabilità dei decreti-legge, faceva riferimento ad un'antica stagione di questo Paese totalmente superata, che riguardava il fatto che i decreti si susseguissero senza mai avere una conversione in legge. Come si vede, già questo sgombrerebbe il campo da ogni equivoco: non è questa la circostanza, non siamo dinanzi ad un decreto‑legge che non è stato convertito e che viene reiterato attraverso un nuovo decreto‑legge, ma una situazione che è stata regolamentata da una legislazione definita è stata poi successivamente superata da questo provvedimento, che affronta una contingenza, una nuova emergenza, e per di più la disciplina anche diversamente. Se fosse come sostiene il collega D'Alì, cari colleghi, sarebbe sempre vietata la proroga dei termini: tutte le leggi che prorogano i termini sarebbero incostituzionali. Mi rendo conto che addurre un inconveniente non è un argomento, ma la questione principale positiva rimane quella che ho detto:

Non esiste nessuna norma costituzionale che si assumerebbe violata per il fatto che si individuino dei siti predeterminati attraverso un provvedimento legislativo di fonte primaria da partedel Parlamento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'invocazione dell'articolo 120 della Costituzione

quelle condizioni di benessere e quegli *standard* di qualità concernenti appunto i diritti civili e sociali. La nostra Nazione non può accettare che una Regione bella e importante come la Campania versi in una condizione di disastro, non soltanto ambientale ma anche igienico-sanitario, tale da alterare in maniera gravissima le condizioni e la qualità di vita dei cittadini di quella Regione. A questo punto si giustifica pienamente l'articolo 120, che a quella norma dell'articolo 117 fa richiamo, per sostenere che, in caso di inadempimento da parte delle Regioni o degli enti locali,

che anche la censura ricordata, quella di una sorta di violazione dei poteri dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, è invocata non a proposito. La possibilità data al commissario di requisire e utilizzare anche quelle discariche che sono state sequestrate dall'autorità giudiziaria, signor Presidente, ha assolutamente precedenti nel nostro ordinamento indiscutibili. Non ha nulla a che vedere con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, anzi, se mi è consentito esprimere una mia personale opinione, dovremmo tutti cercare di compiere uno sforzo affinché i beni oggetto di sequestro non vengano a deperire durante tutto il periodo del processo, fino a quando non interviene la confisca che li mette definitivamente nelle mani dello Stato.

senza nessuna requisizione. Cito solo le norme in materia di contrabbando, che consentono, dopo il sequestro e prima della confisca, che un bene dello Stato venga messo a disposizione dello Stato medesimo affinché ne faccia uso. Penso si tratti di una norma utile, una norma utile, importante e opportuna e che bene abbia fatto il legislatore a prevederla dal momento che non solo non inficia i poteri di autonomia e di indipendenza della magistratura (che farà il suo corso

come definire tale rapporto, ma il fatto che si utilizzi un bene sequestrato non può essere un argomento e, vivaddio, invocare addirittura l'autonomia e l'indipendenza della magistratura mi sembra in questo caso eccessivo. Le censure fatte dalla 10a Commissione, signor Presidente, sono argomentazioni di puro merito relativamente ai consorzi di bacino. Perquanto riguarda la questione finanziaria,

se non con determinati requisiti, mentre gli altri, invece, possono essere superati in via ordinaria. La Commissione bilancio non ha fatto censure di questo genere e invocare addirittura

mi sembra davvero l'invocazione di un precetto costituzionale che ha inteso tutelare ben altro, cioè la possibilità per gli enti locali di dotarsi di strumenti finanziari appropriati. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco tutte le osservazioni fatte dal collega D'Alì, che sono state oggetto di approfondita discussione

della magistratura, sul fatto che si intervenga all'interno dei poteri degli enti locali, siano talmente destituite di fondamento che non meritano l'accoglimento di quest'Aula.

Questa è la normalità tecnica, ormai consolidata e non da qualche anno, ma da qualche decennio nel nostro Paese ha e probabilmente ormai da un secolo in altri Paesi che da questo punto di vista sono più avanti del nostro. Questo è quello che fanno quasi tutte le Regioni italiane, chi meglio, chi peggio, comunque la normalità è questa. Su questo non c'è da intervenire né da un punto di vista legislativo, perché è già previsto da tempo immemorabile proprio dal punto di vista delle leggi, né da un punto di vista tecnico perché da inventare non c'è più niente; si può solo eventualmente migliorare ulteriormente i processi in atto, ma anche questo fa parte della normalità dello sviluppo tecnologico: ogni volta che si fa un inceneritore o un termovalorizzatore nuovo,

nessuno. Dopo le cose che ho detto in un minuto e mezzo, la domanda che ogni cittadino italiano si pone è la seguente: come mai c'è il problema rifiuti in Campania

tratta di un problema quantitativo. Se più o meno è sempre un chilo al giorno la quantità di rifiuti che i cittadini campani producono,

a mettere a disposizione o discariche autorizzate o termovalorizzatori. Questa cosa evidentemente in Campania per un po' c'è stata, poi le discariche sono andate a esaurimento perché anche per i non addetti ai lavori non è difficile capire che la discarica è un buco che si riempie:

In Campania è successo questo: le discariche prima erano dei buchi, poi sono state riempite, poi sono diventate dei pianori, poi delle collinette, delle colline e delle montagne ed a un certo punto sono finite.

luogo, è certo che non fanno raccolta differenziata e quindi peggiorano il problema perché metà del problema potrebbe essere risolto se la raccolta differenziata fosse fatta;

Perché oggi siamo qui, nel Senato della Repubblica, rappresentanti di 59 milioni di cittadini, a discutere di un problema locale? Non si deve fare una legge nazionale per risolvere un problema locale.

il Presidente della Provincia di Napoli, il Presidente della Regione campana - tutti casualmente della sinistra - e commissariarli, perché sono incapaci di fare il mestiere per cui i cittadini li hanno eletti.

l'anno scorso, all'atto dell'insediamento, promise che in dieci giorni avrebbe risolto il problema rifiuti nelle strade della Campania.

la settimana scorsa Bertolaso e la dottoressa Di Gennaro ci hanno detto che, se non si riapre la discarica di Ariano Irpino che è un completamento, il piano regionale non sta in piedi, vuol dire che sulla Campania non si è fatto niente per sei-otto mesi. Allora sono assolutamente contrario a ridare maggiori poteri a chi in sei-otto mesi non ha risolto il problema. E dato che non siamo qui per fare demagogia, vorrei ricordare a certi professori che il problema della Campania - qualcuno ha riso otto mesi quando l'ho detto - è nazionale, perché i rifiuti presenti in Campania arrivano da tutto il Paese, specialmente dal Nord (e io sono del Nord), da quel Nord che cerca di criminalizzare i cittadini campani e si ricorda solo alla fine che ci sono anche degli amministratori campani, perché forse qualche volta c'è stato insieme. Venendo alle questioni più tecniche, sono convinto che il provvedimento in esame sia pieno di questioni incostituzionali, a partire dall'articolo 1 dove si parla di «deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria».

ripetono giustamente che la magistratura deve essere rispettata. Credo che vada rispettata anche quando difende la tutela dei cittadini. Vorrei sentire la vostra parola su questo.

chi ha amministrato male una Regione, sperperando soldi e soldi, e non solo una Regione, ma anche il commissariato? Infatti, le indagini della magistratura e della Commissione di inchiesta

approvo la posizione del senatore D'Alì e ritengo che tanti amici nel centro-sinistra, che hanno lavorato onestamente e giustamente per difendere la magistratura da certi attacchi anche faziosi, che hanno lavorato con serietà per difendere i cittadini dalle vessazioni verificatesi in alcune situazioni del Paese, dovrebbero oggi alzarsi e a gran voce dire «no» a questo decreto, perché è palesemente incostituzionale.

momenti di incostituzionalità che offre il provvedimento, e in effetti lo ha dimostrato illustrando in maniera rigorosa e assolutamente convincente tutti i punti in cui il provvedimento confligge con la Costituzione. A fronte di questa facilità nell'illustrare l'incostituzionalità, devo rilevare l'imbarazzo del centro-sinistra nel sostenere la costituzionalità del provvedimento, dalle stesse dichiarazioni del senatore Sinisi, che possono essere paragonate ad una escursione sugli specchi, all'assenza del senatore Villone, che solitamente è colui il quale illustra questi provvedimenti con grande precisione e rigore: evidentemente, lo scrupolo di fine studioso e costituzionalista è prevalso sulle necessità politiche e partitiche contingenti del sostenere la costituzionalità. Al di là di queste affermazioni di principio,

che giustificano la questione pregiudiziale di incostituzionalità, ad iniziare, n particolare, dalla reiterazione, cui ha fatto riferimento anche il senatore D'Alì, che vìola in maniera palese il principio secondo il quale i decreti-legge non possono essere reiterati anche se assumono una veste o un contenuto diverso, visto che nella sostanza questo provvedimento pone gli stessi momenti di difficoltà, la stessa normativa, gli stessi poteri e, nel contesto, può essere definito una sorta di fotocopia di precedenti provvedimenti. Oltre a questo, non va dimenticato che la individuazione delle aree di particolare valore paesaggistico ambientale e protette vìola di per sé stesso questo principio; il fatto che debbano essere individuate per essere adibite a discariche o comunque a risolvere i problemi dell'emergenza evidentemente indica un altro momento di criticità.

costretto ad intervenire per far sì che fosse liberata la strada di accesso ad una delle discariche. Ma il motivo più rilevante, forte e scandaloso di preoccupazione è quello relativo alla utilizzabilità e possibilità da parte del commissario di disporre dei siti sequestrati o sottoposti a provvedimenti cautelari da parte dell'autorità giudiziaria. È una palese, scandalosa violazione del principio della divisione dei poteri

Consentire la possibilità da parte del commissario di avvalersi, di disinteressarsi, di non tenere in nessun cale la misura reale adottata dal magistrato, evidentemente evidenzia questa invasione forte, preoccupante del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario, a parte il fatto che questa possibilità concessa al commissario straordinario consente in molti casi di cancellare le tracce del reato; quindi, un procedimento penale instaurato, iniziato su determinati reati, a seguito di questa possibilità scompare nel nulla, si cancella un reato. E questo è un caso nuovo, di scuola, direi, per la sua perversione, per la sua contrarietà a princìpi elementari e fondamentali. Ma vi è di più, Presidente, posto che l'articolo 2, al comma 1 (ultima parte), dà la possibilità al commissario di sottrarre all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato di emergenza un determinato sito. Questo significa che, se in quel momento, da parte del gestore di quel sito, sia esso commissario o autorità delegata, venga commesso un determinato reato contro la salute pubblica o l'ambiente crei un pericolo forte, il magistrato non può intervenire per interrompere quest'azione criminosa. Penso sia la prima volta che si assiste alla emanazione di una norma così stravolgente, confliggente ma in maniera evidente. E questi sono anche i motivi per cui giustifico l'assenza di qualche persona che doveva forse appropriatamente illustrare e sottoporre all'attenzione dell'Assemblea questo momento così pericoloso. Ma, signor Presidente, tutto il provvedimento, così come evidenziato, confligge con la sostanza dell'articolo 120 Il senatore Sinisi contesta proprio questo, ma allora non c'è a questo punto che dare un risvolto politico alla situazione, posto che l'articolo 120 concede la possibilità al Governo di sostituirsi nell'esercizio di alcuni poteri regionali nel momento in cui si creino situazioni di grave emergenza, situazioni atte atte a provocare un pericolo grave per la incolumità, la sicurezza oppure quando lo richiedano altre impellenti ragioni derivate dall'incapacità da parte dell'ente territoriale di gestire una situazione. È questa norma sostanzialmente un atto di accusa contro la gestione emergenziale da parte della Regione Campania

così fallimentare, scandalosa e così costosa, costata allo Stato ben 2 miliardi di euro, senza ottenere alcun risultato, ma facendo sì che questi denari questi denari fossero dissolti in consulenze, in favoritismi, in clientelismi. Ecco, questo è uno dei motivi per cui vi è una sorta di ribellione, di pudore da dover provocare in tutti un rigurgito morale e moralistico, se volete, a far sì che ci si opponga in maniera ferma al fatto che gli stessi organi, le stesse strutture continuino in quella che è stata una dispersione enorme di danaro, ma soprattutto contro quello che ha incrinato un principio morale, proprio della politica nobile, e che ha posto a Napoli, in modo particolare, ma in tutta la Regione Campania, la questione morale da parte di coloro i quali hanno avvertito questa sensibilità e possibilità. Quindi è una norma che, se se fosse costituzionale, comunque costituirebbe un atto di accusa chiaro, evidente, forte nei confronti di questa gestione. Non dobbiamo, inoltre, dimenticare che tale situazione ci ha posto all'attenzione mondiale in senso negativo. Se prima era stato il «Times» e altri giornali europei ad evidenziare questa situazione, è stata questa scandalosa emergenza ad essere evidenziata dai giornali americani e ieri addirittura dai giornali russi, i quali non riescono a spiegarsi come possa essere accaduto questo. In effetti, è più è più facile far capire ad un non campano il mistero della Trinità, che non la gestione dei rifiuti in Campania. È una gestione che coloro i quali la vivono sulla propria pelle, nell'offesa della propria dignità di uomini, di cittadini e, soprattutto, di politici possono capire e avvertirne tutto il peso.

Per evidenti ragioni di economia, non ripeterò pedissequamente le argomentazioni portate dai colleghi a sostegno della fondatezza di tutte le eccezioni proposte; sembra però che due sottolineature si impongano. La prima, è quella relativa alla sconcertante sovrapposizione e confusione di poteri che si viene a determinare violando l'impalcatura costituzionale. Bene hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto a richiamare l'attenzione dei colleghi parlamentari che sono stati e sono magistrati e che oggi fanno parte dell'attuale maggioranza, in relazione a un provvedimento in forza del quale viene addirittura sospesa l'efficacia di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, determinando evidentemente una situazione di confusione tra i poteri dello Stato assolutamente inammissibile e tale da violare uno dei princìpi cardine del nostro ordinamento costituzionale. La prima sottolineatura era stata oggetto - e bene ha

che non si è limitata, così, «a volo di uccello», a rammentarla, ma ne ha fatto motivo di precisa osservazione alla Commissione di merito, richiamando l'attenzione sulla circostanza che era assolutamente inammissibile, perché costituzionalmente viziato, quel passaggio in forza del quale

Su questo, tra l'altro, in Commissione è stato fatto un approfondito tentativo di riflessione, invitando la maggioranza e il Governo, che apparentemente si è come blindato all'interno di questo testo, a comprendere che, in effetti,

Purtroppo, tutto ciò è rimasto lettera morta, una sorta di dialogo fra sordi. L'ultima fra le sottolineature che portano a non poter che suffragare la fondatezza di questa eccezione

articolo, Presidente, si istituisce un principio in forza del quale viene meno anche il principio della proporzionalità dell'imposizione fiscale e dell'imputabilità, perché a carico degli incolpevoli cittadini campani andrà globalmente anche il costo del risanamento dell'emergenza, violando qualunque norma di carattere fiscale in materia, per come la nostra Costituzione, tra l'altro, le delinea.

violati anche i princìpi che la Costituzione garantisce in materia di equità fiscale. Leggetelo l'articolo 7; i campani lo leggeranno e si renderanno conto di che cosa questo Parlamento si accinge a votare.

nel corso dell'illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità, è stata sollevata, in numerosi interventi di colleghi dell'opposizione, la questione relativa alla corretta copertura del provvedimento. Si è sostenuto, in sostanza, che una delle ragioni per le quali il provvedimento dovrebbe essere considerato contrario alla nostra Costituzione è il fatto che esso vìola, in alcune sue norme importanti, l'articolo 81,

derivano dalle opinioni e dalle posizioni del senatore Morando e non già del presidente della Commissione bilancio. Vorrei far notare ai colleghi e a lei, signor Presidente, che, per quanto i profili di copertura del provvedimento, è necessario partire da una netta distinzione tra due fasi d'intervento tra di loro molto diverse, relative all'emergenza rifiuti in Campania. Vi è una prima fase, quella dell'emergenza (e certamente non sto ad illustrare perché si possa fondatamente ritenere che esista un'emergenza rifiuti in Campania, che mi sembra sufficientemente provato dalle immagini che ognuno di noi ha potuto vedere in televisione nel corso degli ultimi mesi), che pone pone il tema di un intervento di tipo emergenziale e il provvedimento, con grande precisione, assegna tale compito al commissario. Naturalmente questa prima fase d'intervento deve essere finanziata, e a mio giudizio lo è correttamente, a valere su risorse destinate nel bilancio agli interventi di emergenza.

il volume delle risorse necessarie per l'intervento di emergenza in Campania nei prossimi giorni, sotto la gestione diretta del commissario, è disponibile e sufficiente

- la Commissione ed il Governo - hanno assicurato che tutti gli interventi di emergenza sono finanziabili nel quadro del tetto delle risorse fissate per quel che riguarda le disponibilità messe

nell'illustrazione delle pregiudiziali, e cioè che vi siano interventi di emergenza da mettere finanziariamente a carico delle tariffe. È assolutamente vero, invece, che l'articolo 7, dal 1º gennaio 2008, mette la gestione ordinaria

dal 1º gennaio 2008 le tariffe debbano assicurare il pagamento integrale del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti:

- che dal 1º gennaio 2008 realizza per la Campania esattamente la stessa situazione che si realizza per tutti i Comuni e le Regioni d'Italia, compiremmo un intervento di merito assolutamente ultroneo rispetto alle nostre competenze.

ma che ritengo fondata sui fatti): la Commissione bilancio ha condotto un esame approfondito degli aspetti di copertura relativi al provvedimento e ha concluso che sia la gestione dell'emergenza, sia, dal 1º gennaio 2008, quella dell'ordinario servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono finanziariamente coperte in modo corretto. Aggiungo che, a mio avviso, un problema molto serio di profili costituzionali per gli aspetti di copertura si sarebbe posto, paradossalmente,

È per questa ragione che le une e le altre ipotesi sono state considerate dalla Commissione bilancio lesive dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Se ne deduce, paradossalmente, che avremmo determinato - o determineremmo, in questo caso non come Commissione bilancio, ma come Senato - la violazione di un principio costituzionale essenziale anche sotto il profilo fiscale, se sostenessimo, colleghi, che nella Regione Campania

Ciò non accade in alcuna parte d'Italia e a regime è sacrosanto non debba accadere nemmeno in Campania, datosi che, se questo accadesse (cioè se i cittadini della Campania, per una qualche ragione, a regime, dovessero avere il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti per una qualche quota coperto dalla finanza dello Stato centrale), si determinerebbe una grave disparità di trattamento per i cittadini italiani, giacché ci sarebbero cittadini che non debbono farsi carico di oneri che invece sono affrontati da altri cittadini in ogni altra parte d'Italia. Considero che qui si sarebbe determinato un vero *vulnus* costituzionale, ma è vero esattamente l'opposto, se leggiamo il provvedimento. Esso, infatti, punta a gestire l'emergenza, a chiuderla e ad aprire una fase di perfetta omologazione tra i cittadini campani e quelli del resto d'Italia per quel che riguarda

Presidente, ritengo che il senatore Morando avrebbe fatto bene a impegnarsi per una causa più comprensibile ed anche migliore. Guardate Guardate che il provvedimento, in realtà, non è altro che la presa d'atto e la conseguenza normativa di quattro disastri: un disastro ambientale, un disastro finanziario, il disastro della legalità e un disastro politico. Iniziamo dal disastro ambientale. L'emergenza rifiuti in Campania trae origine da una scelta e da una responsabilità che storicamente è soltanto della sinistra,

di tutte le discariche in Campania. Mette in moto quel meccanismo perché sostiene che sulle discariche vi è una sorta di accumulazione primitiva di profitti criminali e quindi, per battere il crimine organizzato, bisogna chiuderle.

collateralismo con la camorra. Questa è la responsabilità storica. Poi c'è un'altra grande menzogna, quella che tenta di far risalire alla presidenza Rastrelli parte della responsabilità di questo disastro. La presidenza Rastrelli, in realtà, vara un piano regionale dei rifiuti che faceva perno su due termovalorizzatori (in un primo momento, sulla provincializzazione dei termovalorizzatori), ma anche qui si scontrò con la proterva opposizione degli ambientalisti della sinistra che accusavano la giunta Rastrelli il progetto napoletano di termovalorizzatori avrebbe provocato un inserimento - anche qui - del crimine organizzato, mentre grandi investimenti per due termovalorizzatori avrebbero impedito questo tipo di infiltrazioni. Ed ecco allora che si avvia quel processo incompiuto, perché poi la sinistra si oppone anche alla realizzazione dei termovalorizzatori: non solo la sinistra ambientalista, ma anche il PDS.

Questo cortocircuito della razionalità politica, amministrativa e gestionale provoca un disastro ambientale. Sette milioni di tonnellate di rifiuti

i cosiddetti siti di stoccaggio. Per trasportare questi sette milioni di tonnellate di rifiuti pressati occorrerebbero 350.000 Tir: immaginate che disastro ambientale. Non solo, ma due termovalorizzatori dovrebbero essere impegnati a tempo pieno per cinque anni:

anche le coscienze che dovevano porsi a garanzia anche giudiziaria. Infatti, ci siamo trovati di fronte ad un sostituto procuratore iperambientalista che in realtà si accompagnava con imprenditori - i fratelli Orsi - camorristi legati al clan dei Casalesi, una famiglia mafiosa tra le più agguerrite della Campania. Inoltre,

dove grazie a questi meccanismi di potere e di corruttela diffusa bene o male il consenso arriva ancora, ma un disastro di credibilità della sinistra complessivamente nel Paese, tant'è vero che Fassino ha affermato che la sconfitta elettorale e in altre aree dell'Italia è stata provocata anche dall'emergenza rifiuti in Campania. Quindi, questa

in Campania ha rafforzato il suo potere sull'emergenza rifiuti, rischia ora di essere sommersa dall'emergenza dell'immondizia.

è che il senatore Novi prova a spargere un po' di terrore in maniera del tutto infondata. Caro senatore Novi, glielo dico adesso, da medico:

se un fattore ambientale è in grado di indurre un incremento di patologie tumorali, questo non si manifesta prima di un certo numero di anni, che è compatibile tra gli otto e i dieci. Dopo Hiroshima, dove c'era l'emergenza nucleare, le prime leucemie e le prime manifestazioni tumorali in maniera diffusa cominciarono a distanza di alcuni anni.

abusiva e illegale, inquinando i famosi laghetti del Casertano o le aree Acerrane. Se i criminali della camorra rubavano i cavi dell'elettricità per ricavarne il rame e nell'area di Calabricito bruciavano i cavi spargendo diossina sul terreno fino ad avere una incidenza di diossina 100.000 volte superiore ai livelli tollerati e le pecore brucavano l'erba di quel territorio e la diossina ricompariva nel latte delle pecore pecore o delle bufale o delle mucche campane, cosa diavolo c'entrano le ecoballe stoccate nei siti di stoccaggio provvisorio? L'emergenza rifiuti in Campania era quella della camorra che utilizzava la propria organizzazione al servizio delle attività imprenditoriali del Nord. Questa è, mi perdoni, la realtà.

fu vinto da un'impresa che non aveva il *know-how* adeguato, come ha rivelato nel tempo, e nonostante il progetto dalla commissione che la Regione aveva insediato fosse stato giudicato tecnicamente inappropriato; dopodiché il progetto prevedeva che fosse il soggetto privato...

il piano prevedeva una cosa del tutto anomala, e cioè che fosse il soggetto privato ad individuare la localizzazione degli impianti da fare. Questo è il grande *vulnus* introdotto da quel piano, e che è stato uno degli argomenti, insieme ad alcune delle affermazioni fatte dal senatore Novi, che non sono del tutto al di fuori dalla realtà. Ma il dato storico è questo. Mi spiace aver utilizzato parte del tempo a me concesso per provare a ripristinare un po' di realtà, perché quella dei tumori legata all'emergenza dei rifiuti solidi urbani è cosa abbastanza lontana dalla verità. L'emergenza rifiuti che ha provocato il problema in Campania è quella dei rifiuti tossici industriali smaltiti illegalmente in quel territorio.

la situazione dello smaltimento rifiuti in Campania, che già in condizioni di base appare caratterizzata da gravissime difficoltà, presenta una fase di acuzie che viene definita con il termine di «emergenza nell'emergenza».

ci si è sostanzialmente illusi di risolvere la questione attraverso un progressivo ampliamento ed incremento dei poteri straordinari affidati ai commissari di turno. Ricordo al riguardo che si sono alternati prefetti, presidenti di Regione, prima il commissario Catenacci e adesso il commissario Bertolaso, in quanto capo della Protezione civile. La realtà si è incaricata di dimostrare l'inefficacia di questo approccio. Nel tempo il Commissariato ha rischiato di diventare una parte del problema più che la soluzione. Quando il costo dello smaltimento esplode nella progressività che si è notata in Campania, è facilmente comprensibile quel che accade. In una recente audizione ci è stato comunicato dal commissario Bertolaso che lo smaltimento di un certo quantitativo di rifiuti aveva richiesto una spesa di 10 milioni di euro a fronte del fatto che ne sarebbero stati sufficienti quattro per attrezzare un impianto di discarica che avrebbe potuto smaltire un quantitativo dieci volte superiore. Quando, in sostanza, il costo dello smaltimento si moltiplica per dieci o per quindici, è evidente che si realizzano degli extraguadagni che vanno ad alimentare soggetti che hanno tutto l'interesse a che l'emergenza rifiuti non abbia fine. L'inefficienza della catena istituzionale campana è chiaramente all'origine di quest'emergenza e non mi sembra che pur nella valutazione, però, della peculiarità della situazione regionale, piagata dal fenomeno dello smaltimento abusivo di rifiuti tossici prevalentemente provenienti da impianti produttivi del Nord del Paese e con la drammatica presenza di una criminalità organizzata fortemente pervasiva che aveva ed ha individuato nello smaltimento dei rifiuti un importante campo di attività e di elevata redditività. In questo senso, anche una legislazione in cui il reato ambientale ha la caratteristica di contravvenzione costituisce un apparato di contrasto legislativo del tutto inadeguato a contrastare un fenomeno che ha quell'elevata redditività di cui si è parlato. Ma anche in presenza di queste specificità, non si può non riconoscere, come già detto, l'inefficienza della filiera istituzionale.

Ci si è opposti sostanzialmente a tutto, non solo ai termovalorizzatori, ma anche a discariche, ad impianti di trattamento, di selezione, di trasferenza e perfino di compostaggio. Va riconosciuto però che negli ultimi anni alcuni fenomeni di proteste locali hanno anche il loro fondamento nel fatto che i siti verso i quali ci i siti verso i quali ci si approccia in casi di emergenza continuano ad essere sistematicamente gli stessi e quindi tornano i nomi di Ariano Irpino o di Parapoti, che hanno già pagato un prezzo eccessivamente alto rispetto a questa emergenza.

Pur dette queste cose, noi riteniamo che nel decreto ci sia una possibilità di avviare una fase reale di uscita dall'emergenza grazie anche al coinvolgimento dei Presidenti di Provincia, che mostrano una nuova sensibilità: infatti, a Salerno, a Benevento, ad Avellino fioccano le proposte per ospitare impianti ed individuare siti perché tutti ci si rende conto dell'ulteriore non sostenibilità del fenomeno che sta provocando danni gravissimi all'immagine della Campania, ma anche alla sua economia. economia. Immagino che un turista che vede quelle immagini sui giornali di tutto il mondo non voglia trascorrere le proprie vacanze in Campania o che un imprenditore non voglia fare investimenti in un territorio con quelle criticità. Questo decreto, con tutte le sue

Presidente, ho chiesto di avere l'elenco degli iscritti a parlare, che di norma dovrebbe essere già stato definito nella serata di ieri. Le chiedo la cortesia di farmi avere questo elenco, in maniera che si possa avere certezza sulla prosecuzione dei nostri lavori di oggi e di martedì prossimo.

perché è un provvedimento normativo che individua i siti da destinare a discarica ed è il commissario delegato ad avere il potere di individuare - cito testualmente dall'articolo 2 - «le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle Il commissario straordinario può agire in deroga ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria; inoltre, alcuni poteri attribuiti ai prefetti della Campania sono particolari perché sono molto discrezionali per assicurare la piena effettività degli interventi su *input* del commissario. Questa è la prima ispirazione. La seconda ispirazione è di sfida, è il tentativo di uscire dalla fase della necessità, è il tentativo di dare alle istituzioni campane un credito, una fiducia per aprire la fase della possibilità:

perché su sua proposta il commissario delegato può revocare la dichiarazione di stato di emergenza anche a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica. Il vero problema e la vera sfida, però, stanno nell'articolo 9.

sia ritirato il vecchio Piano regionale di gestione dei rifiuti e sia adottato il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la Regione Campania. Qui entrano in carico molti problemi perché l'articolo 9 assegna alle Province compiti specifici di individuazione degli smaltimenti, degli impianti, delle discariche, delle cave, degli impianti di CDR e anche delle possibilità di completare l'utilizzazione dei termovalorizzatori. È del tutto evidente che l'ordinarietà prevista dalla prima parte del decreto si sposa e determina la possibilità prevista nell'articolo 9. Se non c'è un credibile piano entro tre mesi, la stessa ordinarietà crolla. Se non funzionano i termovalorizzatori, se non sono messe in sicurezza le cave, se non ci sono gli strumenti per il compostaggio, se non si sa che cosa fare del CDR vero e di quello meno vero;

affluenza di risorse sarà dovuta - come, ad esempio, si valutava nella Commissione bicamerale sui rifiuti - ai fondi di sviluppo regionale europeo, al fondo aree sottoutilizzate, a risorse nazionali di cofinanziamento. Se non è così, il tutto non si tiene. Se non è così, non si sa dove mettere i rifiuti ordinari, non si sa come trattare il CDR, non si riesce a costruire e a mettere in funzionamento i termovalorizzatori. Se non è così, riprende la spirale impazzita degli ultimi anni. il collega Morando - è la questione della totale sostenibilità a carico della comunità campana e dell'insieme dell'operazione, della possibilità di attivare fondi europei e fondi nazionali ma in tempo utile, coerente e sincrono e sincrono che dà credibilità o meno a tutta l'operazione. È la questione che dà anche sostenibilità nazionale a tutta l'operazione. Per questo motivo - a parere nostro - occorre un migliore approfondimento della sostenibilità finanziaria prevista

*(DCA-PRI-MPA)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi senatori, con questo decreto‑legge il Governo ha posto il sigillo ufficiale a quella che è stata nell'ultimo decennio l'assoluta inefficienza e la pessima gestione, da parte di Bassolino e delle Giunte di centro-sinistra, dello smaltimento dei rifiuti solidi della Regione Campania, cioè del disastro ecologico più imponente degli ultimi decenni. Ancora una volta ci troviamo in presenza di un provvedimento che, con interventi straordinari, dovrebbe far superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania e dovrebbe garantire l'esercizio dei propri poteri poteri agli enti ordinariamente competenti. Ma come è possibile, signor Presidente, che si possa superare l'emergenza proponendo e approvando norme che, senza il coinvolgimento degli enti locali, possano essere corroborate per il perfezionamento del piano dei rifiuti? Come è possibile, signor Presidente, che si possono individuare i siti per le discariche provinciali scegliendo in alcuni casi parchi o aree naturalistiche oppure cave abbandonate, anche sottoposte a sequestro giudiziario? Ma come è possibile che i Verdi, gli ambientalisti e il ministro Pecoraro Scanio abbiano potuto avallare questo ulteriore disastro ecologico? Certamente con il loro silenzio sottoscrivono ancora una volta il loro attaccamento alle poltrone e al potere a tutti i costi. Ma come è possibile, signor Presidente, pensare che un piano per un'emergenza così importante possa essere portato a compimento senza aggravio di spesa? Ma il Governo lo sa che il superamento dell'emergenza richiede una combinazione di varie misure come l'utilizzo delle discariche, il compostaggio e il riciclaggio di rifiuti, la realizzazione di un combustibile da rifiuti di qualità nonché l'impiego degli impianti di termovalorizzazione? In parole povere, signor Presidente, come si può realizzare e portare a compimento il piano di smaltimento dei rifiuti solidi senza un vero e proprio piano rifiuti? Signor Presidente, per chi abita a Napoli, per i campani, devo evidenziare in questa sede, perché gli italiani lo sappiano, qual è la presa in giro che viene effettuata dall'amministrazione regionale di Bassolino e dall'amministrazione comunale di Napoli della Iervolino nei confronti di tutti i cittadini della Campania.

di come si amministra la cosa pubblica a Napoli, di come si tiene conto della vita, effettiva e sostanziale, dei napoletani e dei campani,

ho cercato di portare un contributo sulla base del pensiero federalista che mi contraddistingue nel mondo della politica. È da tempo che fuori dal Palazzo si parla con ferocia contro il mondo della politica e i comportamenti dei politici. Per di più, 15 giorni fa, per lavoro, sono dovuto andare a Napoli e posso dire di essere rimasto fortemente impressionato per quel che ho colto

poteva essere redatto diversamente, poteva essere riscritto o poteva anche non arrivare qui, dato che continuo a non capire, sempre per il mio spirito federalista,

e qui il mio pensiero va ai ragazzi di Napoli, che vivono anche in mezzo alle strade e che devono sopportare una situazione di indecenza nel rapporto con la politica della propria città.

un senatore della Repubblica che non dimentica che nello stadio di Napoli era stato affisso uno striscione con la scritta «Bossi crepa». Non lo dimenticherò mai, ma la mia coscienza cristiana e cattolica mi dice di andare incontro ad emergenze che vergognosamente sono a discapito di tutta la nostra classe politica

di tutti - che a piene voci criticava il nostro mondo, dicendo che la politica è nel caos e non riesce a risolvere i problemi del Paese.

di primavera di una politica, dove ci sono dei problemi che riguardano non la salvaguardia del Governo che - sono il primo a dirlo - deve andare a casa, ma quei bisogni

cultura ecologica. Nel decreto parliamo anche di raccolta differenziata. Sono pienamente convinto che la raccolta differenziata non la si possa fare per decreto.

sacchi di immondizia: quello verde per il vetro, quello giallo per la carta, quello rosso per la plastica, il bidone per l'umido eccetera. Non sono cose che si possono inventare per decreto.

di gestione di questo momento di emergenza della città, che non possiamo dimenticare. Come politici, non possiamo fare

e sicuramente al di fuori del palazzo continuerebbero a dire che la politica è impotente anche nelle questioni che riguardano le persone. che riguardano le persone. Occorre in particolar modo guardare anche a quella parte dell'elettorato che non può esprimere ancora il suo giudizio con un voto e che deve subire un disastro amministrativo che va condannato.

che si ricorra a una legge dello Stato per stabilire, Comune per Comune, i siti delle discariche di immondizia e i siti di quei Comuni dove le discariche sono precluse. Se vogliamo dirla tutta, non è nemmeno normale, signor rappresentante del Governo, che ad occuparsi in prima persona di tale questione debba essere il Presidente del Consiglio e che un decreto‑legge in materia ambientale non porti la firma del Ministro dell'ambiente. La sola giustificazione plausibile è che nell'emergenza sulla quale interviene questo ennesimo decreto di normale non c'è più nulla. Il decreto sfiora appena la gravità di un'emergenza a tempo indefinito che a volte viene richiamata anche nel testo con allusioni rassegnate. Come all'articolo 2, dove si incarica il commissario delegato di individuare le soluzioni - si fa per dire - ottimali per «l'eventuale» (qui la cautela è d'obbligo) «smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione», che ammontano ormai a milioni di tonnellate di cui non si sa cosa fare, salvo continuare a buttare soldi nel costo degli stoccaggi. Intervengo, signor Presidente, soltanto per toccare una questione, una sola, che è oggetto costante di interdizione politica e che riguarda l'incenerimento dei rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, nei casi in cui si procede a differenziarla e anche nei casi in cui esiste quantomeno una forma di raccolta. Degli inceneritori capaci di recupero energetico, gli innominabili termovalorizzatori, è interdetto anche il nome: ad esempio, la Regione Campania ha approvato, in data recentissima, un ponderoso *corpus* legislativo che disciplina in ogni particolare il futuro desiderabile di una Campania a rifiuti zero.

i signori senatori mi permettano di mettere a confronto la condizione ambientale della Campania - quale tragicamente conosciamo - con quella dell'Emilia quale ci è stata descritta, pochi giorni fa,

informato che l'Emilia produce circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti urbani l'anno, ne ricicla circa il 40 per cento con la raccolta differenziata

Questi inceneritori non sono ubicati in contrade irraggiungibili e remote; quello di Bologna è a una decina di chilometri dal centro della città, mentre quello di Forlì è a quattro chilometri. Cosa ne risulta circa la qualità dell'ambiente e dell'atmosfera? La situazione emiliana per l'opera di questi otto termovalorizzatori - o inceneritori che dir si voglia - è forse peggiore di quella campana? Gli *standard* di presenze turistiche delle coste emiliane e romagnole sono forse danneggiate rispetto a quelle della Campania dove - a quanto si dice - quest'anno c'è una vera e propria caduta delle prenotazioni turistiche per effetto degli degli spettacoli mediatici derivanti dai rifiuti lasciati in mezzo alla strada? La produzione alimentare dell'Emilia con punti di eccellenza che circolano per il mondo è forse inferiore a quella di una Campania dove non si può più produrre la mozzarella e non si possono più mangiare le fragole a rischio di inquinamento di diossina, una diossina presente quando i termovalorizzatori non ci sono ancora?

una cittadinanza che viene offesa ogni giorno nei suoi diritti più elementari. Vorrei sommessamente invitare i colleghi ambientalisti (ne vedo qualcuno in circolazione nell'emiciclo) a considerare quello che a me appare un pregiudizio - sbaglierò nella mia valutazione - non giustificato dal

la Romania ne produce 378 e non ne brucia nessuno. Personalmente spero che la condizione ambientale della Campania riesca, una buon volta, ad avvicinarsi alla Svezia, anziché restare uguale a quella della Romania. Signori senatori, con la fine dell'anno la gestione commissariale avrà termine.

il commissario - sentiti tutti coloro che devono essere sentiti - riesca ad adottare il piano per il ciclo industriale dei rifiuti in Campania, comprensivo di tutta l'impiantistica necessaria che oggi, come abbiamo appena finito di dire, manca del tutto. Comunque, con il nuovo anno, la gestione del ciclo dei rifiuti in Campania non sarà più commissariale e ritornerà alla normalità istituzionale con un accordo di programma - e concludo, signor Presidente - che richiami tutte le che richiami tutte le istituzioni ad assumersi le responsabilità di rispettiva competenza e, come si è soliti dire nel linguaggio corrente, c'è da incrociare le dita, visti i precedenti. Alla fine dell'anno, però, mancano oltre sei mesi, quali il compito di far fronte al disastro resta affidato al commissario, titolare di un'impresa improba, che trova più resistenze critiche ed ostacoli che sostegno proporzionato alla difficoltà dell'impresa.

Occorre un'azione risoluta che non ceda alla disinformazione, alla demagogia, alle resistenze cieche e agli illegalismi palesi. La mia, signor Presidente, non è un'opinione, è una citazione: sono le parole con cui il 22 maggio il presidente Napolitano ha esortato, dovrei dire ammonito, il Governo ad attuare il precedente decreto, gli amministratori locali a non capeggiare contestazioni, i cittadini a non ostacolare le misure indispensabili per evitare il disastro che insieme è economico, ambientale e sanitario, nonché lo Stato

è evidente che la questione della distribuzione dei tempi diventa funzionale per evitare che si continui con questo andamento. Ora, quando vi è un'attività ostruzionistica, il rispetto degli orari del Regolamento deve essere assolutamente rigoroso, al fine di dare certezza all'andamento dei lavori e ai ruoli di maggioranza ed opposizione. Pertanto, cosa accadrà? Martedì pomeriggio l'attività ostruzionistica impedirà il voto del provvedimento, certamente questo slitterà a mercoledì mattina e poi, se il Presidente vorrà concedere ulteriore tempo, magari anche a giovedì, e via discorrendo. Signor Presidente, si tratta di un decreto-legge, che - come sa - avrebbe dovuto essere discusso e approvato dal Senato già nella giornata di ieri, secondo le nostre previsioni regolamentari e l'annuncio della convocazione dell'Assemblea.

(dovrebbe essere un comportamento ordinario, da qui alla fine della sessione di luglio). È bene chiarire subito come stanno le cose, perché altrimenti corriamo il rischio di avere una gestione dei lavori d'Assemblea che

anzitutto le opposizioni, ma anche la maggioranza: vorrei pertanto pregarla, signor Presidente, di fare in modo che tutti e due i ruoli - di maggioranza e di opposizione - siano tutelati nel rispetto degli orari previsti per la seduta, che prevedono appunto la chiusura alle ore 14.

Presidente, dopo aver contattato tutti i Gruppi: è quindi pensabile che il capogruppo del suo Gruppo, senatore Boccia, non glielo abbia comunicato. Credo che il ritardo del decreto-legge sia conseguente non all'ostruzionismo, ma ad un lavoro svolto in Commissione

*(Aut)*. Signor Presidente, esprimo apprezzamento per lo sforzo riassuntivo compiuto dal relatore e riconosco l'impegno profuso da tutta la Commissione per integrare il testo nei suoi numerosi punti di imprecisione.

In premessa, non condivido affatto l'idea che debba essere addirittura il Parlamento nazionale ad indicare puntualmente la localizzazione di discariche, aree di stoccaggio e rispettive esenzioni o alternative. Ancora una volta, abbiamo trasformato la Commissione in una sorta di Consiglio comunale o regionale alternativo a quelli legittimati e obbligati, a mio avviso, in merito. Il Parlamento si trova caricato di una responsabilità per la quale è impossibile invocare la sussidiarietà. Mi sembrano ovvie alcune considerazioni, intorno alle quali, però, si fatica a trovare un riscontro di sistema nel testo. È certo, per esempio, che chi produce rifiuti li deve anche smaltire. È certo che i costi di una gestione ordinaria devono essere totalmente coperti dalla tariffa (nel testo, peraltro, si parla ancora di TARSU, per di più come fosse una novità a venire dopo il primo gennaio prossimo venturo). È certo che qualunque ulteriore intervento straordinario, dopo il fatidico primo gennaio 2008, dovrebbe avere costi a carico del bilancio della Regione Campania. È certo che, nella attuale emergenza, i poteri del commissario o ci sono, e sono tutelati dallo Stato nel loro esercizio, o non ci sono, e allora vanno integrati in quanto tali e non sostituendo il Parlamento al commissario (che, dopo un decreto come questo, dovrebbe essere esautorato dal suo compito, nonostante egli stesso possa averlo indotto, per coprire ulteriormente il proprio agire). Vorrei, poi, capire - tra l'altro - come l'articolo 4 possa "coerenziarsi" con il disegno di legge n. 772 sui servizi pubblici locali. Delle due l'una: o si elimina l'articolo 4 o si emenda il disegno di legge n. 772 per tutto il resto d'Italia, secondo quanto proposto per la Campania in materia di raccolta differenziata e indifferenziata. Grande preoccupazione desta la previsione dell'articolo 2, con riferimento ai rapporti della gestione commissariale con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per tutte queste considerazioni sembra infine assurdo che si possa passare da una gestione straordinaria ad una ordinaria, come il testo del decreto prevede, in brevissima prospettiva. Dobbiamo ragionevolmente e istituzionalmente prendere atto della circostanza, palesata nelle numerose audizioni in Commissione, della incomunicabilità fra commissario, Regione, Province, Comuni: nessuno di questi livelli sembra in grado di impostare atteggiamenti utili per passare da un "oggi" di emergenza a un "domani" di normalità. E non si parla mai di camorra, che è il convitato di pietra a questo tavolo. Per tutelare la dignità dello Stato, credo sarebbe molto più opportuno che il Governo operasse con decisione tramite il commissario, che ha già poteri (e deve avere anche la forza per esercitarli) in base alle norme vigenti. Se lo Stato vuole o deve intervenire, lo faccia sino in fondo, ciascun livello istituzionale esercitando i propri poteri: individuare i singoli siti, in questo senso, non mi pare compito né del Parlamento nazionale, né (spero di poterlo dire) del Presidente della Repubblica. Il commissario ha un ruolo e poteri: se del caso, li possiamo integrare, ma non possiamo sostituirci a lui. Questi poteri il commissario li deve esercitare; meglio, li deve poter esercitare e in questa precisazione sta il grave compito dello Stato, oggi - forse - carente. Li eserciti, dunque, o rinunci all'incarico. Comprendo perfettamente l'emergenza, ma non credo sia possibile che in quest'Aula si scarichino le mille contraddizioni di quelle istituzioni locali (nonché talune incomunicabilità interne al Governo nazionale), coinvolgendo il Parlamento - a mio avviso - oltre il necessario. Ribadisco la mia personale difficoltà a sostenere la conversione in legge di questo decreto-legge. nuova finestra") *(FI)*. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, dopo oltre 13 anni di inarrestabile emergenza rifiuti in Campania e lo sperpero di quasi 2.000 miliardi di vecchie lire, come ha ricordato il senatore Novi, con finanziamenti dello Stato a fondo perduto, ci ritroviamo drammaticamente ingigantito lo stesso problema. Benché sia tristemente nota l'endemica complessità sociale e territoriale in questo settore è doveroso rimarcare e stigmatizzare le responsabilità politiche, regionali e locali, e ben si sa chi chi ha governato e governi in questi luoghi. I contenuti del disegno di legge, stranamente non firmato da un Ministro dell'ambiente impareggiabile campione del non fare, infischiandosi del danno economico che procura all'Italia (come nel caso di termovalorizzatori, TAV, Ponte sullo Stretto, centrali elettriche di ogni tipo, perfino idroelettriche), ma bene attento a non disturbare i delfini e il passo di cicogne e quaglie, dimostrano del fallimento di alcuni capisaldi della visione velleitariamente ecoambientalista del Governo e soprattutto del Ministro che lo condiziona laddove, articolo uno comma nel disegno di legge si impongono interventi in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico‑territoriali, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico‑sanitarie si sospendono provvedimenti di sequestro di siti da parte dell'autorità giudiziaria. Mi sorge spontanea l'ironia, a fronte delle dichiarazioni del Ministro e dei suoi ambientalisti per esempio nel rispetto del cosiddetto principio di precauzione sbandierato in convegni e simposi per casi ove il temuto danno ambientale, di salute, e quant'altro non è neppure dichiarato dal mondo scientifico, come per esempio l'inquinamento elettromagnetico, per poi tranquillamente approvare le deroghe sopra ricordate,

non totalmente in linea con alcuni colleghi della mia parte politica, sono favorevole in varie parti al disegno di legge, specie per quanto attiene ai riferimento ai poteri e alle deleghe del commissario nominato, al quale anche in Commissione ho espresso solidarietà e fiducia per avere accettato l'arduo compito. Mi preoccupa che, anche questa volta, i politici regionali e comunali possano nascondere le loro responsabilità dietro l'operato del commissario, ma contemporaneamente non siano favorevoli a taluni poteri a lui stesso attribuiti. Alcuni vincoli disposti dal disegno di legge non non mi trovano totalmente d'accordo: per esempio, l'obbligo di utilizzare i consorzi (articolo 4), pure con il potere di accorpamento o scioglimento (comma 3); velleitario l'articolo 8, che prevede che non devono derivare nuovi oneri a carico dello Stato. Stato. Vorrei però rimarcare che il disegno di legge sembra non tener conto dei numeri, che sono l'essenza vera dell'emergenza in Campania. Il Governo indica quattro siti da utilizzare come discarica: a parte i problemi di incompatibilità territoriale (confinanza con aree protette), ben note sia per la stampa, sia per manifestazioni incomprensibili (anche per la partecipazione di esponenti politici aventi il dovere di risolvere e non creare problemi), ricordo che c'è stato l'impegno per l'ordine pubblico di oltre 800 operatori di polizia per vari mesi

Il primo, considerato nel disegno di legge, è l'emergenza relativa ai rifiuti nuovi e recenti, quelli sparsi per le strade o mal depositati senza trattamento in luoghi assolutamente

i quattro siti potranno contenere al massimo 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti, il che significa che a fine 2007 la capacità residua sarà di 1,5 milioni di tonnellate che potrà servire forse fino al 2008 per la quantità dei rifiuti solidi Dove andranno i 7 milioni di tonnellate? È quindi irrinunciabile una forte sinergia tra tutti i sistemi di smaltimento, partendo dalla raccolta differenziata,

al trasporto quotidiano già esistente, altri 350.000 camion, ciascuno con 20 tonnellate di rifiuti, avranno ingloriosamente percorso le strade, purtroppo non solo campane, alla ricerca di improbabili luoghi di smaltimento.

sul fatto che numerose interrogazioni parlamentari presentate, alcune delle quali proprio su questa materia, non hanno trovato ancora risposta.

il numero dei presenti visto che né la televisione SKY né Radio radicale quando trasmettono le sedute del Parlamento consentono a chi ci ascolta di prendere nota di questo non poco rilevante aspetto che caratterizza i lavori parlamentari. Ebbene, il Governo Prodi, che ha battuto ogni record della storia per numero di Ministri, vice Ministri e Sottosegretari, si presenta nel rapporto con il Parlamento in modo arrogante, saccente e presuntuoso, come abbiamo avuto modo di verificare anche dallo sguardo, tra l'ironico e l'offensivo, del ministro Padoa-Schioppa nella recente esperienza sulla "telenovela" Visco, trattata in quest'Aula. E dunque, vedere che un tale numero di Ministri, vice Ministri e Sottosegretari non si prende cura di rispettare una delle prime prerogative dei parlamentari, quella che fa riferimento alle azioni di sindacato ispettivo, qualifica come non mai questo Governo. E non aggiungo altro, per carità di Patria. Venendo ora all'esame del provvedimento in questione, vorrei innanzitutto sottolineare che in Campania non si parla più di emergenza rifiuti. Siamo oramai da anni alla catastrofe dei rifiuti e tutto ciò è stato determinato da un malgoverno consentito il termine - malavitoso della Regione Campania che è sotto gli occhi di tutti. Ne conosciamo gli sperperi, sappiamo quanto è costato e sappiamo che molti esponenti,

È un provvedimento che, dal mio punto di vista, presenta rilievi di incostituzionalità che comunque quest'Aula poche ore fa non ha voluto riconoscere. Contiene, tra l'altro, alcuni aspetti assurdi. Mi riferisco in particolare

che l'articolo 4, che obbliga i Comuni alla raccolta attraverso i consorzi di bacino, è assolutamente da rivedere. Si tratta di dichiarazioni rese a verbale ed incluse anche nel parere che, come Commissione, abbiamo licenziato. Ebbene, in Commissione ambiente altri esponenti dello stesso raggruppamento Verdi-Comunisti Italiani non hanno voluto sentire ragioni e quindi alcuni emendamenti presentati sono stati respinti.

Iervolino. In questa situazione è francamente difficile prendere la parola e dire qualcosa di significativo. La situazione è così

Mai santo fu più improvvido, considerato che Santa Lucia è la santa protettrice dei ciechi. Sfortunatamente i ciechi politici sono esclusi dalla protezione visti i risultati.

ma è quello di pensare «Facci sognare» che possano d'un colpo scomparire il governatore e il Sindaco di Napoli che sono fra i principali artefici di questo disastro ambientale. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

l'11 febbraio 1994 era la data della prima ordinanza commissariale con la quale si delegava il prefetto di Napoli quale commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania; è prevista la cessazione dello stato di emergenza, almeno così prevede il disegno di legge all'esame dell'Aula: 14 anni di gestione commissariale che coincidono con 14 anni di fallimenti. 14 anni di fallimenti che meritavano da questo decreto e da questo disegno di legge ben altra risposta risposta e ben altro coraggio da parte del Governo e della maggioranza nel prefigurare una via chiara di uscita dall'emergenza. 14 anni di sprechi, inefficienza, poca trasparenza; 14 anni che hanno visto bruciare 2 miliardi di euro e che hanno visto dall'altro lato un aggravamento dello stato emergenziale. aggravamento dello stato emergenziale perché nulla è cambiato in materia di politica dello smaltimento: lo sversamento in discarica politica con la quale si affrontò la prima emergenza del 1994, lo stesso sversamento in discarica è la soluzione proposta oggi con il disegno di legge all'esame dell'Aula per affrontare l'ultima emergenza in ordine di tempo. un forte aggravamento e una variante inusuale nel metodo di individuazione dei siti da adibire a discarica. un forte aggravamento perché 14 anni di politica dello sversamento hanno comportato di fatto l'esaurimento in Campania delle volumetrie disponibili. Parlo di esaurimento delle volumetrie disponibili in Campania perché sin dal primo commissariamento, quello del 1994, tutto i commissari che si sono succeduti nel tempo hanno

Ricorrendo sempre ai soliti siti si sono esaurite le volumetrie disponibili per questa strategia di smaltimento. Quando qualche volta si è pensato o si pensa ancora di ricorrere a qualche nuova e originale individuazione, originale individuazione, queste hanno finito o finiscono comunque con l'interessare aree limitrofe alle discariche già esistenti e utilizzate sin dal 1994.

Se questi siti verranno tutti e due utilizzati, alla fine avremo un intero territorio trasformato in una vera e propria pattumiera.

sola variante. La variante consiste - come dicevamo - nella modalità di individuazione dei siti, modalità di individuazione che passa dalla titolarità del commissario delegato al Parlamento. Con questo disegno di legge, se approvato, di fatto non si capisce quale ruolo debba svolgere il commissario appunto commissariato da questo Parlamento. L'intervento del Parlamento nell'individuazione dei siti deriva dal fatto che, non avendo più il commissario delegato la forza di imporre i soliti siti, l'onere di individuare i siti di discarica passa al Parlamento il quale, dal momento che alcuni dei siti da sempre utilizzati sono sotto sequestro giudiziario (uno per tutti Difesa Grande), votando questo disegno di legge autorizza addirittura il commissario delegato ad utilizzare le solite discariche, anche se nel frattempo sono state sottoposte a provvedimenti giudiziari. Presidente, colleghi, è fallita l'attuazione del ciclo integrato in Campania e ci dobbiamo interrogare sul perché è fallito entrando nel merito, perché dobbiamo dire le cose fino in fondo: non realizzati, 7 CDR che - ormai è dimostrato - non producono combustibile per i termovalorizzatori; li possiamo chiamare rifiuti aggiungendoci qualche aggettivo (rifiuto nobile), li mettiamo in ecoballe, casomai li sistemiamo diversamente dai rifiuti solidi, ma sono qualcosa di diverso dal dal combustibile che può essere bruciato nei termovalorizzatori, i quali ultimi comunque non ci sono. Il ciclo integrato è fallito anche togliamo l'anche - soprattutto per l'infiltrazione mafiosa e camorristica, infiltrazione favorita da un regime commissariale che si è protratto per così lungo tempo. Un regime commissariale di così lunga durata porta inevitabilmente, oltre alla istituzionalizzazione del commissariamento che non pensa più forse a svolgere i propri compiti ma semplicemente ad autosostenersi nel tempo,

quando le norme dello stesso sono in buona parte o quasi totalmente in contrasto con un piano regionale, quello della Campania, che non è stato preso in alcuna considerazione dal Governo. Per questo motivo voteremo contro il provvedimento. Non ci saremmo aspettati, da questo decreto, la solita proroga al 31 dicembre, perché al 31 dicembre 2007 farà seguito il 31 dicembre 2008; ci aspettavamo pochi mesi, con il coinvolgimento del territorio, ed un disegno che ci avrebbe portati alla gestione ordinaria. Questo non è, non c'è stato il coraggio, non c'è stata la determinazione, continueremo con le fasi emergenziali e per questa ragione il nostro voto sul provvedimento

non è notizia di oggi, ma data da un tempo lungo almeno quanto l'abbandono al degrado e al sottosviluppo di Napoli e del Mezzogiorno. Fin dal secondo dopoguerra, le discariche campane sono state oggetto di attenzioni e collusioni da parte della camorra e nessuna istituzione o amministrazione fino ad oggi è stata in grado di risolvere il problema. Si è tenuta incancrenita una situazione in cui si sottraggono miliardi di euro allo Stato, ai cittadini, alla sanità, ai servizi sociali, alle politiche occupazionali per un servizio che non è un servizio e che produce profitti enormi solo per chi con l'emergenza ci guadagna. È di aprile la relazione della Corte dei conti che parla di un *flop* per i rifiuti con la gestione dei commissari al Sud di 1,8 miliardi: 400 milioni solo per stipendi e sede. È impietosa l'analisi sulle gestioni commissariali della Corte dei conti, ma oggettiva; descrive un sistema che ha messo l'emergenza nelle mani di imprese pubbliche o società miste pubblico-private spesso non competitive, inefficienti, polverizzate, in un intreccio difficilmente districabile tra interessi pubblici e privati. Ancora, la Corte dei conti sostiene che la gestione commissariale, attribuendo competenze straordinarie agli organi ordinari (perché il più delle volte sono stati gli stessi Presidenti di Regione a rivestire la funzione di commissario), ha creato un circolo vizioso perfetto in cui l'inefficienza del regime commissariale ha assicurato a sé stesso la sopravvivenza. Mentre i commissari si impegnavano a sopravvivere, in tutte le Regioni interessate la produzione dei rifiuti è aumentata, la raccolta differenziata è rimasta al palo e i limiti minimi fissati dalla legge - vorrei ricordare che la finanziaria sogna

I progetti sono rimasti sulla carta, i poteri speciali sono stati usati soprattutto per affidare il servizio aggirando i vincoli di gara in contesti ambientali - cito testualmente - «difficili per la presenza di una radicata criminalità economica». Per di più, agli operatori è stata spesso data carta bianca su tutte le decisioni fondamentali, con il risultato che, priva del cappello dell'autorità pubblica e dell'accordo con le comunità, ogni iniziativa è incappata nelle barricate delle popolazioni, spesso spalleggiate dagli amministratori locali per motivi elettorali. Risultati che fanno a pugni con la montagna di risorse impiegate e gestite, secondo i magistrati, in un intreccio perverso fra sciatteria amministrativa, assenza di controlli e gestione allegra di stipendi e consulenze. E tutto questo è, fra l'altro, accaduto anche perché le varie autorità centrali

afferma che non esiste soluzione di continuità tra il ciclo dei rifiuti smaltiti legalmente e la camorra, che detiene interamente il *business*. I rifiuti sono il nuovo oro per la camorra, che ha deciso di investire tutto su questo anziché sul traffico di droga, perché ci sono meno rischi e i guadagni sono maggiori. I rischi sono minori perché le organizzazioni criminali di stampo mafioso godono delle complicità di imprenditori e di amministratori senza scrupoli. Ebbene, di fronte a questa analisi impietosa ed oggettiva, io credo che il problema che andiamo ad affrontare non possa e non sarà certamente risolto dalla conversione del presente decreto. Per fare un salto di qualità sul fronte della gestione dei rifiuti, non basta una soluzione tecnica e tanto meno legislativa.

occorre la vigilanza delle autorità centrali, occorre il coinvolgimento delle popolazioni nelle scelte più delicate. Ho difficoltà per questo a sostenere la conversione di questo decreto-legge, anche perché ho appena di cui do lettura - e qui concludo il mio intervento ringraziando il Presidente che mi dà la possibilità di spendere qualche secondo in più - secondo cui oggi è accaduto ad Avellino che, al grido di «Buffone, vattene via», centinaia di persone hanno circondato e colpito con calci e pugni l'auto del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, Guido Bertolaso, giunto ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, per proporre agli amministratori e alle associazioni ambientaliste la possibilità di riaprire la discarica di Difesa Grande. Il corteo di auto è stato bloccato dai manifestanti in Piazza Plebiscito.

Signor Presidente, ho chiesto la parola sull'argomento da ultimo trattato dalla senatrice Rubinato, cioè della vicenda che ha visto coinvolto il commissario Bertolaso ad Ariano Irpino, che mi dà l'occasione evidentemente di esprimere tutta la solidarietà al commissario straordinario, ma anche di segnalare e di inquadrare questo episodio all'interno di una vicenda più complessiva e, soprattutto, rispetto ad un'area, in particolare quella di Ariano Irpino, che da troppo tempo

la discarica per anni e che oggi si ritrovano di fronte ad una soluzione, la più semplice e ovvia possibile, della riapertura della discarica stessa. È evidente che questo, nonostante il grande senso di responsabilità delle istituzioni e della popolazione locale, può determinare qualche problema e qualche difficoltà. Vorrei che si tenesse conto complessivamente di questo dato e di questo contesto e a maggior ragione ci sentissimo responsabilizzati nel dibattito su questo decreto e sugli interventi che esso prevede, che a volte rappresentano un'inutile forzatura rispetto ad alcune comunità reazioni che non si possono certo giustificare e tanto meno condividere, ma che vanno inquadrate all'interno di questo contesto che determina grandi difficoltà. Tra l'altro aggiungo, solo per informazione doverosa, che la vicenda si è sviluppata in questi termini: era previsto un Consiglio comunale aperto, quindi l'amministrazione locale aveva accolto l'invito del prefetto a determinare le condizioni per un confronto con il commissario Bertolaso ad Ariano Irpino - ripeto -con un Consiglio comunale aperto; purtroppo, questo Consiglio comunale aperto non si è tenuto proprio per il clima che si era creato e che, in un certo qual modo, era anche presumibile. Allora concludo in questo modo: modo: nessuna giustificazione ad atti di intemperanza e di violenza; nessuna giustificazione a qualsiasi scelta di deresponsabilizzazione; tuttavia qui sta emergendo un dato che non riguarda il commissario Bertolaso, che fa quel che può: il dato è che non si può ritrarre la politica dall'assunzione di responsabilità rispetto a questo problema. Oltre all'episodio spiacevole, credo che questo sia l'elemento che emerge con grande forza e che ci richiama tutti a una grande responsabilità, che non può cadere sulle spalle di Bertolaso o di qualsiasi altro commissario o funzionario pubblico.

Bertolaso e sottolineare che comunque l'istituzione territoriale, il Comune appunto, su sollecitazione del prefetto, aveva organizzato un Consiglio comunale aperto, Bertolaso voleva entrare nel merito delle problematiche. Bisogna che il Parlamento si faccia carico di questo nuovo caso e che rifletta su tutta la materia dell'emergenza rifiuti in Campania, in particolare sull'individuazione dei siti che verrebbero ad essere utilizzati senza una conoscenza specifica dei vari territori. Morra. Dicevo prima che ovviamente la Presidenza non entra nel merito delle valutazioni politiche rispetto a tutta questa materia, anche se di certo non possiamo che stigmatizzare tutti gli atti di violenza che si compiono, che in ogni modo non trovano alcuna motivazione e giustificazione. Mi sembra molto corretto che noi si prosegua il nostro lavoro, perché siamo impegnati a dare una soluzione, che l'Aula dovrà

Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, queste brutte notizie allarmano perché creano un ulteriore clima di preoccupazione, perfino di disagio. Penso che occorrerebbe invece ritornare a costruire tutti insieme un clima di distensione e di serenità, perché ne va della credibilità complessiva delle istituzioni. qui oggi a discutere il terzo decreto speciale in due anni per la Campania; francamente, avremmo voluto farne a meno, perché dal febbraio del 1994, l'anno della prima dichiarazione dell'emergenza, ad ora sono passati ben e dopo tutto questo tempo non può esserci più nulla di straordinario. Del resto, la permanenza in carica di un commissario straordinario è la conferma di un segnale di grave sofferenza. L'emergenza ancora una volta non è stata risolta e l'obiettivo categorico di riconsegnare il potere di decisione agli organismi democratici è nuovamente posticipato nel tempo. La prima osservazione che viene da fare è che alla scadenza del 31 dicembre 2007, prevista dal precedente decreto, data in cui scadrà la nomina del commissario straordinario, occorrerà un cronoprogramma che accompagni e preceda tutte le azioni che si decide di compiere; un cronoprogramma chiaro, fattibile, credibile (come si è anche chiesto direttamente al commissario durante la sua audizione), dove le scadenze siano frutto di concertazione con gli enti locali e di intese con la popolazione, che è sempre più allarmata ed esasperata, come abbiamo visto dai brutti avvenimenti

Per dare credibilità al processo per uscire da questa interminabile fase di crisi è necessario che chi governa la Regione Campania si dia da fare, torni ad essere un protagonista, per sollecitare ad essere un protagonista, per sollecitare una data finale certa e improrogabile di approvazione di un nuovo piano regionale dei rifiuti. Questo è importante perché non è pensabile immaginare che, fissata una scadenza, scatti un'ora «x» che faccia immediatamente e automaticamente

un ruolo di riferimento istituzionale e politico che dia fiducia a chi effettivamente in questo periodo ha molto sofferto. D'altronde, alcuni segnali vanno nella giusta direzione. La recente approvazione della legge regionale sui rifiuti della Regione Campania, che ha indicato la costituzione degli ATO per quando si tornerà a regime,

Dopo il fallimento del piano Rastrelli, che è stato ricordato semplicemente come una misura utile per la soluzione dei problemi della Campania (ma così non è stato), sappiamo tutto sulla produzione e sui costi dei rifiuti e sulle tecnologie che dovrebbero essere adottate. Sappiamo molto sulle ecomafie e sul pericolo che c'è nell'intreccio fra queste ultime e la gestione dello smaltimento dei rifiuti. Sappiamo di una delicata situazione in cui vari interessi si scontrano anche fuori dalla legalità. Basta ricordare un dato che è stato ampiamente citato: quando il costo per lo smaltimento dei rifiuti passa in pochi anni da 14-15 euro a tonnellata a 140‑160 euro a tonnellata, ci sono tutte le premesse e le condizioni affinché il malaffare si possa approfittare di questi facili guadagni. A questo punto occorre tornare a decidere democraticamente, a rimettere nelle mani dei Comuni, delle Province e delle Regioni ciò che un commissario non può fare, ma può solo aiutare a fare: questo deve essere il suo ruolo. Certo, non possiamo ignorare le responsabilità politiche di chi, in questi 13 anni di commissariamento, non ha saputo evitare l'incancrenirsi della situazione, dovuta essenzialmente al grave errore iniziale, del 1996, datato al piano Rastrelli, quello di avere consegnato alla FIBE del gruppo Impregilo l'appalto unico nella costruzione di sette impianti di CDR e di un impianto di termovalorizzazione per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. un piano che ignorava l'impegno per la raccolta differenziata e per una gestione integrata dei rifiuti e che, nonostante le opposizioni e i richiami (anche da parte del Ministero dell'ambiente di allora), non è stato mai fermato.

e gli impianti, che dovevano essere il fulcro del sistema di smaltimento dei rifiuti, declassati da produttori di CDR, cioè da combustibile per termovalorizzatori, a frazione secca, e la FOS (frazione organica stabilizzata) declassata a semplice frazione umida da porre in discarica.

Peggio ancora, nascono interrogativi sull'utilizzazione del delicato sito di Terzigno, collocato nel Parco nazionale del Vesuvio, in mancanza di un prodotto compatibile con quell'ambiente

alcuni mesi fa tra il presidente del Parco e lo stesso commissario al fine di intervenire nell'ambito dello stesso Parco attraverso una ricomposizione riqualificata ambientale delle cave e delle discariche, utilizzando esclusivamente del FOS. Per tutto questo siamo preoccupati, ma siamo anche responsabilmente impegnati a trovare le migliori soluzioni per uscire dall'emergenza in atto che, autorevolmente, il Presidente della Repubblica ha definito tragica, ponendola così all'attenzione di tutta l'opinione pubblica nazionale, delle forze politiche e del Parlamento. Il Parlamento è oggi chiamato, in definitiva, a decidere ciò che non è stato possibile decidere localmente.

Ci ha convinto il fatto che tale scelta è accompagnata da un buon lavoro preparatorio della struttura del Commissariato, nonché dalla presentazione poi, da parte del Ministero dell'ambiente, di relazioni tecniche con l'obiettivo, per

oltre naturalmente alla sicurezza degli impianti, alla salute dei cittadini, all'inquinamento del territorio e delle falde acquifere che saranno salvaguardate. Le correzioni apportate in Commissione, che sono state sostenute dai Gruppi parlamentari dell'Unione e che, per certi aspetti, hanno trovato anche un conforto da parte dei colleghi della minoranza, hanno delineato un risposta ai tanti interrogativi iniziali che riguardavano, innanzitutto, il rafforzamento del ruolo delle Province attraverso l'istituzione dei subcommissari,

di una contabilità che sappia distinguere i costi sostenuti, in modo tale che gli abitanti della Campania, al pari degli abitanti di tutto il resto del Paese, possano pagare la TARSU o la TIA solo per il servizio effettivamente ricevuto.

È un provvedimento non solo inutile, ma controproducente che amplia e non restringe la crisi dei rifiuti in Campania e rivela, purtroppo, una sintonia di fondo tra le pessime scelte della Giunta Bassolino e quelle del Governo Prodi. Prodi. In Campania l'emergenza c'è ed è gravissima, ma questo decreto la esaspera ed è destinato - questa purtroppo è la mia previsione - a trasformare l'emergenza rifiuti in un'emergenza di ordine pubblico e le notizie che arrivano da Ariano Irpino confermano tale preoccupazione. Quello di Ariano, un Comune importante della mia Provincia e dell'Irpinia, è un caso che va studiato con attenzione e di cui parlerò fra poco. I motivi di un giudizio così negativo sono molti e complessi: il principale è che questo decreto non rappresenta alcuna inversione di tendenza rispetto al passato e non cambia alcunché rispetto a quello che lo ha preceduto pochi mesi fa. In quell'occasione espressi voto contrario, differenziandomi dal Gruppo dell'UDC, che invece aveva aperto una linea di credito, astenendosi. Oggi, l'orientamento contrario di tutto il Gruppo testimonia, purtroppo, che le mie preoccupazioni erano fondate e che nemmeno l'intervento di Bertolaso - ridotto a fare la foglia di fico dell'irresponsabile gestione Bassolino - è servito a cambiare le cose. Il dato politico più importante è che il decreto non risolve, ma cronicizza l'emergenza rifiuti: il clima in Campania è esplosivo. Ieri abbiamo letto addirittura, con grandissima preoccupazione, che i vigili del fuoco di Napoli, a fine turno, vengono sottoposti ad un processo di decontaminazione, come in un film di fantascienza. Inoltre, le evidenze epidemiologiche illustrate ieri in Commissione, qui al Senato, testimoniano dati raccapriccianti sull'aumento delle malformazioni neonatali, dei tumori e dell'inquinamento ambientale della Campania. Il presidente Bassolino passerà alla storia come il responsabile di un arretramento pauroso della qualità della vita nella Regione, avendola portata agli ultimi posti in Europa. Infatti, non vi è solo l'emergenza rifiuti, ma anche quella sanitaria, occupazionale e criminale: la Campania, un tempo definita Regione *felix*, oggi fa il giro del mondo Altro dato assolutamente negativo del decreto è l'insistenza su una politica che si è rivelata fallimentare: quella delle discariche. La conduzione dell'emergenza rifiuti può essere efficacemente raffigurata come l'atteggiamento della massaia che cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto: il problema, però, è che l'altissima densità di popolazione della Regione rende impossibile nascondere sotto il tappeto‑discarica tonnellate di polvere. È proprio questo - cioè la sproporzione tra i rifiuti prodotti e quelli smaltiti che ha mandato in tilt, ormai da decenni, il sistema in Campania e qui sta la responsabilità politica e morale del centro-sinistra che ha amministrato la Regione negli ultimi quindici anni: aver ignorato l'evidenza e chiuso gli occhi di fronte alla realtà, omettendo di realizzare un piano organico di uscita dalla crisi. Regione e commissariato hanno rinunciato al proprio dovere d'indirizzo, ed è questa una colpa grave: vedere che oggi questa scriteriata linea di condotta viene avallata e sostenuta anche dal Governo nazionale rende tutto più difficile. Quando ci si interroga sul perché delle reazioni delle comunità locali - come quella verificatasi questa mattina ad Ariano Irpino alla riapertura delle discariche - vi è più di una risposta: l'esasperazione, la legittima reazione a inganni e malgoverno e, soprattutto, la certezza di essere governati da una classe dirigente che per quindici anni non è stata in grado di affrontare e risolvere il problema problema alla radice. Le popolazioni della Campania hanno sempre dimostrato, nella loro storia, solidarietà e spirito di sacrificio: se oggi non ne possono più, è perché si sentono giustamente prese in giro da un potere politico che si è preoccupato di sperperare milioni di euro per realizzare le Notti bianche a Napoli piuttosto che togliere i cumuli di rifiuti che che ne ostruiscono le strade. Oggi si pagano la miopia e l'incompetenza - e forse qualcos'altro - della classe dirigente del centro‑sinistra, che cerca di scaricare sugli altri le proprie responsabilità. De Mita, uno dei due diarchi della Regione, in una recente intervista a «Il Mattino», ha dichiarato che non è il momento di ricercare le responsabilità: invece, io dico che solo la ricerca e l'identificazione di queste possono costituire la premessa per uscire dalla crisi, altrimenti irreversibile. È troppo comodo, oggi, invocare solidarietà generiche: dov'era l'onorevole De Mita quando il centro-destra - e non solo, per la verità proponeva di affrontare in altro modo la crisi dei rifiuti in Campania? Dov'era il suo alleato Bassolino, quando l'UDC chiedeva nella Regione di recuperare il piano rifiuti della Giunta Rastrelli, attraverso la realizzazione di una serie di termovalorizzatori,

una crisi di sfiducia, prima che tecnica; una crisi di valori, che sta allontanando i cittadini dalle istituzioni locali. In Campania - lo ribadisco - la situazione è esplosiva e chi la conosce può confermarlo. Voglio ricordare, in proposito, le parole del sindaco di Montecorvino

Questo è il clima di sfiducia in cui si muove la Campania, un clima che il decreto oggi all'esame del Senato contribuirà ad accrescere, perché - come ho ricordato poc'anzi - una politica dei rifiuti basata solo sui piani-discariche avrà due effetti: la non soluzione del problema e l'esasperazione delle comunità locali. È questa la ragione principale della nostra - lo sanno anche i bambini - non possono essere accumulati, ma devono essere distrutti. Ed era, quindi, logico programmare una filiera che cominciasse con la raccolta differenziata e si concludesse con la realizzazione dei termovalorizzatori. In quindici anni tutto questo si poteva e si doveva fare; quindici anni - nell'Europa comunitaria e nel mondo civilizzato - sono un tempo sufficiente per risolvere il problema rifiuti di una intera Nazione. E invece quindici anni, nella Campania di Bassolino, Iervolino e De Mita non sono bastati, non dico per risolvere il problema, ma nemmeno per avviarlo a soluzione. I rifiuti in Campania non li hanno portati gli alieni, il loro accumulo è il risultato di scelte politiche scellerate che hanno precise paternità, scelte che, fortunatamente, cittadini ed elettori della Campania cominciano ad attribuire ai veri responsabili. Chi ha sbagliato, finalmente, comincia a pagare; chi ha pensato di autoassolversi o addirittura di attribuire ad altri le proprie responsabilità, oggi sa che il tentativo è fallito e che il re è nudo. Altro punto debole del decreto è lo stesso che ha impedito finora la soluzione del problema: per sintetizzare, la mancanza di una *exit strategy*. Quando si chiede ad una popolazione di sopportare sacrifici - il che determina la reazione violenta delle comunità locali per essere credibili bisogna dire quanto dureranno i sacrifici, quando finiranno, e come si uscirà dall'emergenza. È questa la condizione per coinvolgere e responsabilizzare e responsabilizzare amministrazioni e comunità locali. Ed è esattamente questo, invece, che manca nella filosofia del decreto, che rende vana ogni prospettiva di soluzione del problema. Con una battuta, direi che noi cattolici siamo inclini al perdono, ma il perdono, per essere tale, deve essere accompagnato dalla coscienza del peccato commesso e da un pentimento sincero. E a noi pare che nessun segnale di pentimento sia emerso in tutti questi anni all'interno della classe dirigente che ha provocato il disastro rifiuti, così come nessun serio segnale di inversione di tendenza e nessuna presa di coscienza della gravità della situazione sono contenuti in questo decreto. Altro punto fondamentale che non convince è l'impostazione del rapporto con le amministrazioni e le popolazioni locali. Né il governo regionale, né il commissariato né i governi provinciali - che sono tutti in mano al centro-sinistra - hanno saputo dialogare e concertare con le comunità locali per identificare i siti delle discariche: attraverso un irresponsabile scaricabarile, si è cercato al contrario di utilizzare un principio di autorità, salvo poi scappare (come è successo a Bertolaso) dinanzi alle inevitabili reazioni dell'opinione pubblica. I vertici regionali e provinciali sono stati soltanto in grado di scaricare sulle comunità locali il peso della crisi. Il Senato deve sapere che il presidente della Provincia di Avellino, l'*ex* onorevole De Simone, dopo un esame lungo, complesso e costoso, all'interno di una apposita Commissione creata all'interno della Provincia, ha proposto a Bertolaso, come discarica per l'Irpinia, un'area, nel Comune di Savignano, classificata da un organismo pubblico per il controllo del territorio come franosa: vale a dire, una discarica in un'area franosa. È davvero un atto privo di qualunque logica, tragico negli effetti, ma ridicolo nella premessa: un atto che ci trasforma in una barzelletta agli occhi dell'Europa.

colleghi senatori giuristi della sinistra, se sia, cioè, possibile scavalcare e sterilizzare iniziative e decisioni dell'unico potere dello Stato - quello giudiziario che in molte aree della Campania, si oppone con coraggio e determinazione all'illegalità diffusa e alle infiltrazioni della camorra nella gestione del ciclo dei rifiuti. A nostro giudizio è un atteggiamento irresponsabile, che non può essere in alcun modo avallato. Questo elemento costituisce un'ulteriore, gravissima ombra sulle scelte del Governo nazionale e di quello regionale e, in conseguenza, anche su quello che è contenuto nel decreto all'esame del Senato. In Campania oggi c'è un'anomalia in più, che non può essere sottovalutata e che questo decreto non corregge affatto: il rapporto tra attività della camorra e gestione del ciclo dei rifiuti. Voglio essere chiaro: la sinistra, con sforzi che apprezzo, si è sempre battuta contro la criminalità organizzata ed ha anche pagato per questo un tributo di sangue; però in Campania questa però in Campania questa stessa sinistra, che definisco finto ambientalista, impedendo da quindici anni la realizzazione di termovalorizzatori e quindi la soluzione definitiva del problema, ha di fatto, anche se in modo involontario, creato le condizioni oggettive perché la camorra si infiltrasse in questo tipo di in questo tipo di movimento economico. Quindi, c'è una contraddizione in termini sulla quale prego i colleghi di riflettere. Se si vuole combattere la criminalità sul piano tecnico occorre impedire che la gestione del territorio, delle cave e delle discariche sia parzialmente ed indirettamente nelle mani della camorra: questo è un punto fondamentale e può avvenire soltanto attraverso la realizzazione di termovalorizzatori che portino a compimento il ciclo dei rifiuti, altrimenti la camorra avrà sempre la capacità di infiltrarsi, come dimostrano purtroppo le indagini giudiziarie che a Caserta hanno portato all'arresto del vice di Bertolaso. I cittadini, le amministrazioni e le comunità locali della Regione Campania, a cominciare da quella di Ariano, sappiano di poter contare in questo quadro sul sostegno e la solidarietà dell'UDC nella difesa dei propri diritti e nella tutela di una dignità di vita che oggi viene loro negata. Per il nostro partito l'emergenza rifiuti in Campania è questione nazionale e come tale deve essere affrontata, trattata e divulgata.

che centinaia di cittadine e di cittadini europei, non solo italiani,

in grave dubbio la correttezza, il comportamento, la responsabilità della catena di comando che ha gestito l'ordine pubblico, pertanto credo sia urgente una Commissione d'inchiesta che attribuisca le responsabilità, che faccia luce su quanto avvenuto, e quindi restituisca alle forze dell'ordine quell'onorabilità che è stata infangata in quei giorni. La fotografia mi ha particolarmente toccato: è quella di Lena, una ragazza tedesca: è stata raggiunta da tre energumeni in divisa, le hanno sfondato il torace a calci, è stata in coma a lungo, fortunatamente si è salvata. Ricordo anche la sua deposizione al processo (processo che non viene ricordato spesso dai grandi mezzi di informazione): con una lucidità incredibile ha raccontato come, dopo il pestaggio, fosse presa per i capelli e trascinata giù per le scale; ha avuto i polmoni perforati, cercava di riparare le costole e la faccia per non sbattere i denti sui gradini con le mani e c'era ancora qualcuno, sempre in divisa, che picchiava con il manganello sulle sue mani per impedirle di ripararsi. Al processo gli avvocati difensori di quei poliziotti si sono permessi anche degli apprezzamenti poco gentili nei confronti di Lena. Credo che dobbiamo a Lena e a tutti i manifestanti di quei giorni a Genova finalmente una verità riconosciuta. Presidente, la mia richiesta è meno vibrante, ma rientra nelle formalità d'uso. Oggi si è celebrata a Roma l'Assemblea nazionale della Confartigianato. Esattamente un anno fa, nella medesima occasione, presentai un documento con il quale chiedevo che alla denominazione della 10a Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo) venisse aggiunto anche la parola "artigianato"; questo perché ce ne occupiamo di fatto, inevitabilmente, ogni giorno e per riconoscere il ruolo e l'importanza di tale categoria: oltre 4 milioni di imprese e circa 15 milioni di addetti. Non ho ottenuto risposta da un anno ed io che sono un indomabile utopista, sebbene mi sia stato detto che è più facile cambiare un Governo che la denominazione di una